Ho passato l'intera mattinata qui al mio posto, ho ascoltato la discussione e ho partecipato a tutte le votazioni. Il caso vuole che a una di esse risulti che io non abbia partecipato: in particolare, la votazione segreta relativa alla richiesta di dimissioni del senatore Giaretta. Io, Presidente, ho sicuramente votato, ho visto anche la luce accesa; non so cosa sia successo. Ritengo vi sia stato un errore, probabilmente ho votato in anticipo o in ritardo. Mi auguro tuttavia che non vi sia un problema anche tecnico, il che sarebbe più serio; infatti, l'errore umano è rimediabile, mentre sull'errore tecnico bisogna intervenire. In ogni caso, Presidente, ciò che a me interessa è che sia dato atto e resti a verbale che ho sicuramente votato;

tutti sanno che sono straordinariamente diligente nel seguire le indicazioni del mio Gruppo e se dissento, come talvolta può capitare, manifesto pubblicamente il mio dissenso. Vorrei, pertanto, che si prendesse atto di ciò.

Signor Presidente, non occorrono molte parole, perché si tratta di riprodurre la Commissione che già nella legislatura passata era stata istituita e ha lavorato. Quando ho iniziato la mia vita politica, molti anni fa, sentivo dire che quando non si sa come risolvere un problema si nomina una Commissione; non ho mai avuto, però, propensione per questo scetticismo. Nel caso specifico, mi sembra che la Commissione, presieduta dal nostro collega Pianetta, abbia lavorato bene e che i problemi, vecchi e anche nuovi, in materia di diritti umani richiedano tutta la nostra attenzione e il nostro impegno.

*(Ulivo)*. Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, desidero esprimere innanzitutto la mia convinta adesione sia al contenuto sia alla parte deliberativa della mozione per l'istituzione di una Commissione speciale sui diritti umani. Non può esistere alcun dubbio in ordine al fatto che il rispetto per l'uomo, per la persona i diritti di ogni individuo siano ormai una conquista e un patrimonio dell'umanità. Non esistono però diritti e, soprattutto, non hanno senso se rimangono privi di tutela, se non esistono sistemi e meccanismi giuridici in grado di garantire l'effettività del diritto stesso. Il diritto di una persona non ha alcun senso se non è garantito sul piano della realtà giuridica quotidiana. In questo ambito, ma ancor più in un ambito internazionale, assume fondamentale, anzi, preliminare rilievo, la conoscenza delle varie situazioni di fatto che teoricamente possono non prevedere, in origine e normativamente, la tutela di un diritto della persona, oppure prevedere tale diritto in astratto ma, di fatto, non consentirne l'esplicazione e, quindi, la tutela. Ben venga, quindi, la costituzione di una Commissione permanente per i diritti umani, proprio ai fini di garanzia e tutela indicati. Mi sia consentito però un breve cenno a due questioni che ritengo molto importanti

la prima questione, bastano poche parole, perché, se da una parte va accolta con estremo favore e, anzi, fortemente appoggiata l'attività del Tribunale penale internazionale,

dall'altra, preso atto delle forti, fortissime resistenze che incontra la piena e autonoma attività di tale organismo, va sottolineata la necessità di un impegno e di un'azione precisa per estendere il più possibile il numero dei Paesi ratificanti la Convenzione istitutiva del Tribunale penale internazionale, pur sapendo bene quali siano gli Stati che non l'hanno ratificata e probabilmente non hanno intenzione di ratificarla per motivi altrettanto noti e sicuramente non nobilissimi. Per quanto attiene alla seconda questione, relativa all'istituzione di una Corte internazionale per i crimini in materia ambientale, non mi nascondo le difficoltà che sono, per certi versi, ancora maggiori rispetto a quelle concernenti il Tribunale penale internazionale. Peraltro, nella situazione mondiale attuale, per di più a pochi giorni dal dal gravissimo allarme lanciato a Parigi da scienziati e ricercatori di tutto il mondo, ritengo ancora più importante muoversi lungo questa strada. Dirò di più, perché da anni esistono e lavorano anche alacremente in tale ottica, enti, istituti e organizzazioni in tutto il mondo. Anche poche settimane fa, da Venezia è partita una convincente e motivata proposta per l'istituzione di una Corte internazionale per i crimini ambientali a opera dell'IAES, l'Accademia internazionale di scienze ambientali, di cui fanno parte alcuni premi Nobel e di cui è presidente onorario il premio Nobel Perez Esquivel. Orbene, se non ci si rende conto e non ci si convince che la questione ambientale ormai ha a che fare con la persona, con i diritti della persona, della collettività collettività e anche delle generazioni future, non si fa cosa utile a noi stessi e alle nostre istituzioni. Il concetto di ambiente ha ormai assunto una connotazione più ampia rispetto al passato e ha a che fare con l'uomo nei suo aspetti essenziali. Per questo ritengo che la Commissione istituenda dovrà tenere conto anche degli aspetti e dei temi che ho testé trattato. È per questo infine che, ribadendo l'appoggio convinto alla mozione avente come primo firmatario

unisco volentieri il mio nome, la mia voce e persuasione a quella del senatore Andreotti e degli altri firmatari della mozione perché ritengo che colmi una lacuna e che ci dia uno strumento particolarmente prezioso in un momento, come quello attuale, di incertezze e di imprecisioni anche tra Stati, anche all'interno delle stesse alleanze, anche nelle stesse parti del mondo e anche al di là delle divisioni che contrappongono parti avverse del mondo. Il tema dei diritti umani, infatti,

Probabilmente nel mondo moderno, che noi conosciamo e nel quale viviamo, la prima definizione formale dei diritti umani si ritrova nei *Federalist Papers* che hanno dato vita alla Costituzione americana. È allora quasi inevitabile ricordare che

della sacralità della persona, nei concetti di delitto, uccisione e parricidio nei quali si identifica l'individuo e non lo Stato come fondamento dell'ordinamento giuridico: è curioso che tale riconoscimento avvenga così presto nelle Carte federaliste alla base della formazione della Costituzione americana. Da allora, Da allora, il seme dei diritti umani è cresciuto all'interno delle Costituzioni degli ordinamenti democratici, anche se è tutt'altro che un diritto al sicuro o un fatto certo ed inconfutabile,

il tribunale locale aveva riconosciuto il diritto di uguaglianza, già garantito dalla Costituzione. Ebbene, quello è un giorno di grande importanza per decifrare certi aspetti della vita e della storia americana. Quel giorno, infatti, il Ministro della giustizia di quel Paese, Robert Kennedy, telefona al Governatore dell'Alabama, imponendogli un *aut aut*: o lo Stato dell'Alabama esce dall'Unione o il nero James Meredith entra nell'università,

dell'ordinamento americano. George Wallace ha dovuto cedere sulla base del fatto che il diritto di una persona veniva riconosciuto come più importante del diritto non solo di uno Stato, ma dello stesso Stato federale e del rapporto tra Stato federale e Stato dell'Alabama. Credo sia un esempio da ricordare quando ci metteremo al lavoro, e spero di poter partecipare a questo lavoro.

nell'Aula del Senato della Repubblica italiana: in questo momento, donne e bambini, che cercano acqua nei pozzi delle aree del Sud del Sudan, sono aggrediti, violentati, oggetto di violenze fisiche spaventose e semplicemente perché si può fare, semplicemente perché la comunità internazionale ha permesso che si faccia, semplicemente perché la comunità internazionale tace. tace. Se istituiremo quest'organo, esso farà in modo che il nostro Paese e la nostra struttura politica, ma anche la nostra opinione pubblica, non si diano pace fino a quando situazioni di quel genere continueranno a ripetersi.

che avrebbe voluto restare e vivere in Italia e che è stata, invece, rinviata nel suo Paese, dove era stata vittima di oltraggio e di violenza,

di una situazione piccola rispetto al Darfur e rispetto al contrasto fra lo Stato dell'Alabama e lo Stato federale americano; si tratta una piccola persona di dieci anni, che ha chiesto al sistema giuridico e statuale di un Paese contemporaneo che il suo diritto venisse rispettato. Ciò non è avvenuto ed io non posso che sperare, con tutto il cuore, che l'esistenza di un organo quale una Commissione sui diritti umani serva per capire, per penetrare, per avvicinarsi, per sapere, per informare, per motivare l'opinione pubblica e per diventare un organo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sottoscritto, a nome del Gruppo dell'UDC, la mozione presentata in questa Camera sulla questione dei diritti umani nel nostro Paese e a livello internazionale. La costituzione di una Commissione del Senato su un problema di così ampio respiro, che caratterizza la fisionomia del nostro Paese e dà un codice genetico molto chiaro alle iniziative di carattere politico, è un'iniziativa che nobilita e sottolinea l'aspetto di una italianità che nel mondo raccoglie consensi. Ma per parlare più nello specifico dei diritti umani, credo vi sia bisogno

casualmente il precedente Governo ha portato avanti la diplomazia preventiva, vecchia intuizione di un Segretario delle Nazioni Unite negli

noi lo abbiamo fatto anche perché la diplomazia preventiva è un aspetto di politica estera che può essere adottato soltanto da Governi animati da valori.

Con l'azzeramento del debito, con la riconversione del debito dei Paesi in via di sviluppo, noi abbiamo improntato una caratteristica tutta italiana. Lo abbiamo fatto non solo in Africa, ma anche in America Latina e in altri Paesi dimostrando, nella difesa dei diritti umani, che non sono soltanto diritti di un modello di società, ma anche diritti per rimettere la persona al centro delle nostre politiche, e ciò sottolinea questa nostra grande e straordinaria vocazione. Quindi, quando ci troviamo oggi a parlare di ricostituire una Commissione che, tra l'altro, ha avuto efficacia anche in precedenza, ci troviamo a trattare proprio questo aspetto; una grande e straordinaria occasione che abbiamo per far sì che anche nelle guerre dimenticate, gli organismi internazionali possano incidere. Ma i diritti umani, cari colleghi, non sono soltanto legati ai Paesi in via di sviluppo, alla diplomazia preventiva, alla politica estera. I diritti umani sono anche la difesa di quei diritti elementari, che vengono violati anche nel nostro Paese. oggi, ascoltando osservatori della politica che si rifanno e si richiamano alla difesa dei diritti umani sui problemi relativi alla giustizia, al sociale, riscontriamo le tante ingiustizie presenti nel nostro Paese.

se possiamo attuare, indipendentemente dal *Club* di Parigi, ulteriori iniziative per la riconversione del debito dei Paesi in via di sviluppo, per il sostegno delle politiche multilaterali con le Nazioni Unite, sostenere quelle Agenzie che possono dare riscontri nel tentativo di far crescere milioni di bambini con più aspettative di vita. Allora, credo che su queste linee possiamo sviluppare un ragionamento forte; possiamo da oggi ripartire, in questa legislatura, non solo nella difesa di tutti quei diritti, ma anche in una lotta forte contro la pena di morte nel mondo. mondo. Credo sia una barbarie consentire, in un Paese che guarda alla globalizzazione con gli occhi del futuro, ad una Europa, soprattutto, che deve diventare interlocutore per evitarla, che in molti Paesi ancora viga di fatto la pena di morte. Dobbiamo lottare perché tutto ciò non possa avvenire, per affidare alle nuove generazioni, non solo di italiani, un mondo più giusto,

indicata nella mozione, di procedere in futuro, come avviene in altri Parlamenti, alla costituzione di un organismo permanente in questa materia. Vorrei pertanto aggiungere solo qualche osservazione affinché affinché l'istituzione di questa Commissione, che io auspico, non sia esclusivamente e soltanto un'affermazione di buona volontà, un'affermazione retorica, ma renda tutti noi consapevoli delle conseguenze politiche e di comportamenti concreti che derivano da un impegno di questo genere sul tema dei diritti umani. La prima osservazione che vorrei fare è la seguente. La centralità della tutela e della promozione dei diritti umani nei rapporti tra Stati comporta una revisione del concetto di sovranità nazionale. Oggi abbiamo uno Statuto delle Nazioni Unite in cui si consente un intervento della comunità internazionale per impedire che un Governo minacci la sicurezza di un altro Stato, ma non si prevede alcuna possibilità di intervento della comunità internazionale quando quel Governo minacci la sicurezza del suo proprio popolo. Quindi, l'elemento diritti umani è sostanzialmente escluso dal novero delle possibilità che le Nazioni Unite assegnano alle decisioni del Consiglio di sicurezza. Pertanto, esso comporta, a mio modo di vedere, forme di limitazione della sovranità nazionale, naturalmente decise dalla comunità stessa e nei modi dei fori multilaterali, e produce anche la necessità di costruire quello che ormai viene definito un vero e proprio diritto dell'ingerenza umanitaria. Non credo che l'impegno degli Stati democratici a difesa dei diritti umani possa prescindere da questa riconsiderazione dei rapporti tra Stati e che possa proseguire mantenendo invece intatta quella concezione della politica estera come *Realpolitik,* che pure ha orientato il comportamento di tutte le democrazie occidentali fino a poco tempo fa, comprese quelle dei Governi italiani, Governi italiani, che in sostanza vuol dire che ogni Paese, ogni Governo, è libero di fare ciò che vuole a casa sua. In secondo luogo, vorrei osservare che il concetto di universalità dei diritti umani, uno dei contenuti più pregnanti della Rivoluzione francese, è stato rivisitato, rivalutato e approfondito più di recente nella parte finale dell'ultimo secolo dal pensiero liberale, anche attraverso la contestazione di quello che viene definito il relativismo culturale. Se si accetta cioè che alcuni popoli, alcune culture, alcuni Paesi, hanno diritto a comportarsi diversamente da noi sul tema dei diritti umani, perché non comprendono la tematica dei diritti umani come noi, si fa un'affermazione di evidente razzismo strisciante. Kennedy diceva che la libertà è indivisibile: se la libertà di un altro essere umano è conculcata, anche la nostra non è piena. Non è un'affermazione da poco questa, perché ci costringe a riconsiderare anche il comportamento che la comunità internazionale ha in materia di intervento umanitario.

così come un passo avanti importante è il senso di colpa che si è impadronito del mondo intero di fronte al mancato intervento umanitario in Ruanda e in Darfur. Aggiungerei anche il ruolo che i *media* stanno assumendo in questa materia, creando forse per la prima volta nella storia dell'umanità una vera e propria opinione pubblica globale,

Quando ci si batte a difesa dei diritti umani è bene non estendere eccessivamente il campo, non creare confusioni, delimitare esattamente quali sono i diritti fondamentali dell'uomo; estendere troppo il campo rischia di rendere meno efficace l'azione di difesa dei diritti umani. Intendo dire che spesso alcuni diritti dell'uomo, come i diritti sociali, il diritto al lavoro, alla previdenza e alla salute, vengono erroneamente inseriti nell'ambito dei diritti fondamentali dell'uomo, con nocumento, secondo me, dell'impegno per la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo. Un'ulteriore osservazione riguarda gli ambiti e i modi di intervento. Credo che dobbiamo considerare l'impegno di questa Commissione che stiamo per istituire

avviene ed è segnalata anche dalla Corte di giustizia europea (penso, per esempio, alla irragionevole durata del processo o alle condizioni penitenziarie in cui vivono alcuni detenuti), e

la condizione delle donne e dei bambini all'interno delle comunità di stranieri che vivono nel nostro Paese. È un problema di dimensioni molto rilevanti e sul quale non possiamo tacere, soprattutto se vogliamo occuparci di analoghe questioni in casa d'altri.

la necessità d'introdurre nel nostro ordinamento (e anche da questo punto di vista la Commissione può avere una funzione di stimolo nei confronti del Parlamento)

perché siamo forse l'unico Paese di civiltà democratica e liberale che non ha una legge che definisca e tuteli sia il diritto d'asilo, attuando fra l'altro l'articolo 10 della Costituzione,

discorso vale anche per i rifugiati che non hanno la possibilità di fuggire all'estero, che è un altro enorme aspetto del problema, spesso non considerato. centinaia di migliaia, milioni di persone che fuggono per paura di vendette e di abusi, ma non hanno la possibilità, i soldi o la fortuna di raggiungere un altro Paese e quindi sono rifugiati all'interno del loro stesso Paese.

La proposta realizzata da diversi

la stessa non diventi una palestra di esercitazione, onorevole senatore Andreotti, di politica estera per alcuni e di discriminazione per altri. I diritti civili e i diritti umani sono stati spesso visti ad intermittenza dal mondo politico italiano, a seconda di chi governasse,

Poc'anzi abbiamo sentito alcune citazioni forbite in un buon dialetto bostoniano dal senatore Colombo,

la facesse da padrone in una Commissione di questo genere, che è l'ambito esatto e preciso, Presidente, dove si possa o essere equi e veramente attenti ai diritti dei bambini, delle famiglie, dei giovani, degli immigrati, degli emigrati e di tutti o fare - ripeto - la classica palestra, dove la demagogia e la retorica possono trionfare sovrane. Siamo stati abituati a questo tipo di demagogia e di retorica ed un caso - lo dico ai miei amici di Alleanza Nazionale, ma lo dico anche al Parlamento - è di questi giorni. I diritti umani sono anche quelli relativi ai diritti alla memoria, di chi non c'è più. In questi giorni abbiamo, con commozione, assistito al programma *Exodus* ed alle grandi manifestazioni, da tutti sentite, in memoria di quello che succedette tra gli anni 1939, 1944 e 1945; però dover, ad esempio, evidenziare - e lo faccio in questa Aula ed é stato oggi fatto dal presidente Fini in una sua nota come un diritto alla memoria di alcuni caduti non sia stato equiparato in questi giorni a quello degli altri. Parlo dei caduti delle foibe, che non sono caduti, non erano combattenti, ma civili italiani

perché i diritti dei bambini palestinesi siano equiparati a quelli dei bambini israeliani, perché i diritti, senatore Colombo,

prenda corpo, perché la stessa, in fretta, venga strutturata dalla Presidenza, perché la stessa cominci a lavorare,

e la FAO, che non possono assolutamente non essere tenuti in debito conto quando andremo ad analizzare i problemi delle discriminazioni, della fame nel mondo e delle libertà individuali.

per motivi istituzionali. Noi contiamo molto sulla possibilità che la Presidenza deleghi qualcuno o vada in prima persona, perché non è giusto dimenticare e non è giusto non essere presenti. Rivado, terminando, al concetto che avevo prima iniziato. Signor Presidente, a lei spetta anche il compito, nella strutturazione di questa Commissione, di un continuo contatto con le scolaresche, con le scuole, con coloro i quali devono forse insegnarci qualcosa. Quindi: promozione di *stage* e corsi di formazione per quei giovani che sui diritti civili molto spesso sono

speranza - ripeto - che il prossimo 10 febbraio anche il diritto alla memoria degli italiani uccisi nelle foibe non rimanga inascoltato dalla Presidenza del Senato.

Signor Presidente, voglio portare il mio compiacimento ai sottoscrittori della Commissione che si dovrà formare e tutta la mia completa adesione. Voglio leggere le prime righe di premessa umani - «si sono recentemente sviluppati, determinando una consapevolezza sempre maggiore in ambito mondiale».

quasi terminando il processo di autoritarismo e iniziando una fase di democratizzazione del Paese. Quello che ho percepito, non solo in Brasile, ma in tutta l'America Latina, dove notoriamente i diritti umani sono stati più volte calpestati, è stato il sentimento pubblico, in quanto la popolazione, non aveva questa coscienza. Ha ragione chi ha scritto che la consapevolezza è abbastanza recente, perché sempre l'argomento principale che si portava avanti era quello secondo cui il fine giustificava i mezzi: i mezzi: per ottenere una pace dal punto di vista dell'ordine, quindi dal punto di vista dello sviluppo dell'attività economica, non importavano, cioè, i diritti umani, che giornalmente venivano violati e calpestati. È molto interessante che in questi anni - l'esperienza è abbastanza lunga, di una trentina di anni - tale consapevolezza sia cresciuta.

e le istituzioni abbiano cominciato ad assumere una maggiore coscienza della necessità della difesa dei diritti umani. Interessante - e questo bisogna metterlo in evidenza nel nostro Senato - è che l'Italia è sempre stata il faro di riferimento dei diritti umani,

il Governo Lula, vi è un'attenzione ancora maggiore. Tale attenzione riguarda, a largo raggio, non solo i diritti politici (basta aprire la stampa brasiliana per rendersi conto della piena libertà democratica che si ha nelle espressioni

(in particolare del Brasile): lo sfruttamento dei minori, la prostituzione, la consapevolezza di ferire dei diritti primari che dovrebbero essere largamente difesi. conclusione, signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare l'importanza di questa Commissione proprio come faro e come punto di riferimento che può avere l'Italia in tutti questi Paesi. Vorrei terminare dicendo: non esportiamo soltanto il *made in Italy*, ma esportiamo i principi dei diritti umani. Faremo un gran bene a tutti i popoli del mondo.

surreale. Chi, nell'Aula di un Parlamento di un Paese democratico, si sentirebbe di dirsi contrario ad ogni iniziativa che possa meglio garantire, difendere ed ampliare sul pianeta i diritti umani? Obiettivamente nessuno. Ma forse non è questo il vero oggetto della nostra discussione. Forse il vero oggetto, che penso animerà la costituenda Commissione e che credo debba animare questo dibattito, è intenderci su cosa siano i diritti umani, da dove vengano le reali minacce ai diritti umani e quali siano quindi i rischi e le opportunità che incontriamo nel

e universale tra la democrazia politica, così come l'abbiamo conosciuta nell'Occidente, e l'affermazione dei diritti umani. Sono in qualche misura gli uni il presupposto dell'altra e senza gli uni l'altra non vive.

‑ di prendere ad oggetto principale delle critiche e degli strali proprio quei Paesi democratici, di democrazia occidentale, i quali hanno posto a fondamento della loro stessa esistenza esattamente l'affermazione di quell'insieme di diritti che va sotto il nome di diritti umani e di dimenticare, invece, che, anche in tempi recenti, le minacce vere e il conculcamento dei diritti umani a livello di massa sono venuti esattamente da quei modelli di organizzazione degli Stati che si sono contrapposti e che hanno combattuto, anche in campo aperto e sul piano della politica internazionale, le democrazie di stampo occidentale.

un certo esito della Seconda guerra mondiale, con l'intervento degli Stati Uniti a liberare i nostri Paesi, noi forse oggi non saremmo qui e non faremmo questa discussione. Se non avessimo visto, qualche decennio più tardi, il crollo dell'altro totalitarismo sotto la pressione politico‑militare delle alleanze occidentali, che in qualche misura oggi vengono messe in discussione - purtroppo - dal nostro Governo e nel nostro Paese, noi non avremmo avuto la possibilità di pensare a difendere e ad estendere i diritti umani. Né sotto il regime fascista e nazista, né sotto quello comunista, infatti, i diritti umani hanno avuto alcuna cittadinanza. Di diritti umani questi regimi hanno fatto strame nella loro attuazione pratica, dando la morte a milioni di persone, solo per il fatto che erano individuati come i nemici

e se qualcuno ha ancora il coraggio di definirsi nazista e se qualcuno ha ancora il coraggio - e sono molti, anche in questo Parlamento - di definirsi comunista, questa lezione della storia, per la quale la democrazia politica di stampo occidentale è il fondamento dei diritti umani, non è stata appresa.

opposizione, che più ha conculcato nella natura stessa dell'espressione di quel regime e nella sua ideologia fondante. Ancora - e non voglio riferirmi allo scorso secolo - da chi viene oggi la minaccia ai diritti umani nel mondo? Non certo dalle democrazie politiche occidentali. occidentali. Dall'11 settembre 2001 abbiamo un nuovo paradigma, per cui abbiamo compreso che la minaccia al modo di vivere, alla libertà, alla democrazia politica e, quindi, alle basi fondanti dell'affermazione dei diritti umani viene da un mondo in cui i diritti umani non esistono in quanto tali, un mondo che ritiene legittimo lapidare, un mondo che ritiene normale mutilare, un mondo che ritiene ordinario conculcare diritti che per noi sono universali e intangibili. Ebbene, rispetto a quel mondo non possiamo porci in una condizione di relativismo culturale ed etico, in base al quale il rispetto della sua libertà sta nell'accettazione supina di questi comportamenti e della vita di comunità che, non solo là,

Allora, se cominciamo ad affrontare questi temi, come spero faremo nella Commissione, ci accorgeremo che la distanza che ci separa anche sul tema dei diritti umani rischia di essere abissale.

in altre situazioni, poco ricorda di quanto è accaduto nella storia e poco dice sul fatto che anche il nostro Paese è venuto meno all'impegno sui diritti umani, per esempio sostenendo la candidatura al Consiglio di sicurezza dell'ONU di un Paese sicuramente totalitario come il Venezuela di Chavez.

americano, ma perché in quel Paese un regime profondamente nemico dell'umanità, quello talibano, è stato sconfitto solo grazie all'intervento militare. Allora dovremmo chiederci anche quanto è necessario l'uso della forza per affermare i diritti umani; quanto è necessario dover venir meno al meglio che possiamo auspicare, cioè un mondo in pace, per non essere in un mondo imbelle di fronte ai terroristi, ai totalitarismi e a chi conculca i diritti umani. In altre parole, se vogliamo affermare i diritti umani, dobbiamo avere delle stelle polari quali la libertà, come l'abbiamo conosciuta in Occidente, la democrazia, così come la conosciamo in Occidente,

organizzata secondo un criterio che non attinge alle democrazie occidentali, fa della pubblica accusa uno strumento di conculcamento dei diritti umani. Numerosi sarebbero i casi che potremmo portare a questo proposito. *(Applausi

per esempio, l'individuazione di un punto di riferimento anche per un'istituzione, che noi abbiamo appoggiato e che esiste a livello locale, come quella dei nostri difensori civici.

organismi nazionali autorevoli e indipendenti - lo sottolineo - per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

e l'Italia tra questi, presumono di garantire già i diritti umani e le libertà fondamentali e quindi di potersi astenere, conseguentemente, dal rafforzare ancora di più la promozione la protezione e dal rispettare i nuovi o i vecchi obblighi sottoscritti a livello internazionale. Penso invece che l'Italia, come qualunque Paese, sia responsabile sia delle violazioni dei diritti universali che avvengono nel suo territorio, di quelli che possono avvenire anche all'estero, a danno sia dei propri cittadini che di quelli stranieri. Esiste il compito anche per noi di migliorare e rafforzare la promozione e la tutela dei diritti umani. L'Italia, come qualunque altro Stato, non è immune dal rischio di violare i diritti fondamentali, né di prevenirne le violazioni. Credo che questo ci riguardi, così come ci riguarda il fatto che l'Italia non abbia una strategia integrata e di lungo periodo sui diritti umani. Vorrei ricordare che il rapporto sul nostro Parlamento, presentato nell'aprile scorso dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, ha avanzato alcune osservazioni in materia: sono stati ricordati alcuni casi in cui la tutela la tutela dei diritti umani nel nostro Paese è *border-line.* Il rapporto fa riferimento alla sospensione dei diritti nei centri di permanenza temporanea, i famosi CPT (che mi pare oggi s'intenda rivedere in modo abbastanza drastico),

per i soggetti arrestati, e non è poco cosa), al fatto che l'Italia ancora non abbia una legge che consideri reato la tortura. A questo proposito, vorrei ricordare un dibattito svoltosi durante la scorsa legislatura alla Camera, di fronte al progetto di legge Pecorella, quando fu presentato dalla Lega un emendamento che considerava la tortura tale solo se reiterata. Ricordo l'intervento, autorevole e appassionato, della nostra attuale Capogruppo Anna Finocchiaro, la quale raccontava di una donna salvadoregna, che lei aveva conosciuto, secondo la quale non erano le torture fisiche quelle che presentavano maggiore sofferenza e che la condizionavano di più, ma il fatto che lei era stata minacciata di subire torture di fronte al proprio figlio. Perché la tortura deve essere reiterata quando è già un abominio?

sancito dall'articolo 10 della Costituzione. L'Italia è l'unico Paese europeo a non aver prodotto una legge organica che lo regolamenti. Solo nel 2005 le richieste d'asilo nel nostro Paese Il programma dell'Unione contempla una legge in materia. Sappiamo che vi sono tre disegni di legge alla Camera e uno al Senato che vogliono affrontare tale materia. Sull'inadempienza in materia di diritto d'asilo, gli ispettori delle Nazioni Unite ci hanno criticato anche parecchio nel loro rapporto e hanno precisato che l'Italia deve dotarsi di una legislazione in materia.

purtroppo, in Italia, sono ancora considerati diritti deboli, spesso di seconda mano, talvolta soltanto enunciazioni di principio

più che la globalizzazione dei mercati e delle merci. Ricorda Cassese che, sebbene sia difficile individuare una Costituzione che vada oltre lo Stato (ce ne rendiamo tutti conto), una una sostanza costituzionale, costituita dalla consacrazione di principi fondamentali, cui è giusto aderire, e e che abbia come fine la tutela dei diritti umani, in realtà oggi è già all'ordine del giorno, perché c'è un grande cambiamento in atto; anche se non se ne vede lo sbocco reale e concreto, è una tendenza a cui moltissimi Paesi sono rivolti.

Signor Presidente, unisco la mia adesione, anche a nome del Gruppo Per le autonomie, alla mozione che ha come primo firmatario il presidente Andreotti. Credo sia molto utile e opportuno dare continuità al lavoro della Commissione sui diritti umani, anche per raccogliere la positiva eredità ed esperienza della Commissione che aveva già lavorato nella passata legislatura con la Presidenza del senatore Pianetta, cui voglio dare atto di aver svolto un grande e positivo lavoro nella passata legislatura. Naturalmente, quando si affrontano tali questioni, si ha l'impressione, soltanto superficiale, che si tratti di temi scontati: non si può non essere d'accordo su un impegno per i diritti umani. In realtà, sappiamo che non è affatto così così e che un impegno serio, che non sia soltanto nominalistico, a favore dei diritti umani comporta una serie di coerenze, nonché la necessità di affrontare nodi assolutamente complessi

Nel codice genetico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è stata la concretizzazione della grande speranza di pace seguita alla Seconda guerra mondiale, questa duplice dimensione è assolutamente evidente: c'è una forte compenetrazione tra l'impegno per la pace, per così dire, la principale ragione sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Carta dei diritti dell'uomo, quindi l'impegno per i diritti umani. Non può esserci vera pace senza rispetto e promozione dei diritti umani. Sembra un'ovvietà, eppure sappiamo come la politica quotidiana, anche nella dimensione delle relazioni internazionali, faccia una grande fatica ad accogliere questo principio. Il governo delle relazioni internazionali, infatti, è in gran parte ancora affidato ad una logica anarchica dei rapporti tra gli Stati e l'idea che debba invece sottostare ad una Costituzione superiore, appunto la Carta fondamentale dei diritti umani, stenta a farsi strada nel mondo. È questa un'utopia tipicamente europea: è stata l'Europa - viene in mente naturalmente la grande lezione di Immanuel Kant, con il suo scritto «Per la pace perpetua» - la culla della della convinzione che la pace possa essere costruita soltanto a partire dall'affermazione di diritti ritenuti primari rispetto alla politica e quindi i diritti umani come il fondamento di una visione della politica internazionale che sottomette i rapporti di forza al diritto internazionale. Si tratta, com'è evidente a tutti, di un'utopia che è ancora assai lontana dell'aver trovato realizzazione, ma proprio per questo impegnare il Parlamento italiano, particolare, a dotarsi di una struttura che rifletta e agisca in questo campo, è un contributo importante, non solo alla causa dei diritti umani, ma anche alla causa della pace. La seconda questione riguarda il fatto che i colleghi che faranno parte della Commissione, e con loro tutto il Senato, dovranno affrontare tre ostacoli formidabili che si frappongono all'affermazione dei diritti umani e che richiedono un impegno tenace e paziente. Il primo ostacolo è rappresentato dal principio della sovranità e della non ingerenza negli affari interni dei singoli Paesi: sappiamo che è uno dei principali fattori che impediscono la messa all'ordine del giorno di problemi che riguardano i diritti umani, la loro difesa ed affermazione. Pensiamo, ad esempio, a quanto sta accadendo proprio in queste settimane all'interno del Consiglio di sicurezza a proposito della Birmania,

anche presenti in Consiglio di sicurezza, ritiene, tuttavia, che il regime birmano non rappresenti di per sé una minaccia alla pace e che dunque non sia immaginabile che il Consiglio di Sicurezza possa occuparsi di quella che viene definita la situazione interna della Birmania. Voi capite che

Nelle relazioni tra gli Stati è del tutto evidente che l'economia ha un grandissimo peso, e non sarò certo io a sposare una visione così ingenua e primitiva dei rapporti internazionali da pensare che l'economia non sia un grande fattore anche di amicizia tra i popoli. Sappiamo, però, che tante volte le ragioni dell'economia sono invocate contro l'affermazione dei diritti umani: si deve chiudere un occhio, in alcuni casi anche tutti e due, sulla violazione dei diritti umani, se non si vogliono perdere

Ecco tre grandi contraddizioni che fanno capire come il lavoro di questa Commissione debba, e possa, essere tutt'altro che scontato. Essa può affrontare alcuni nodi

di una Commissione per i diritti umani a livello internazionale non può non significare anche un impegno del Parlamento italiano, e del Senato in modo particolare, rispetto alle necessarie coerenze a livello nazionale.

Paese assistiamo a ritardi gravi rispetto a *standard* di civiltà che pure a livello internazionale considereremmo assolutamente necessari e scontati. Pensiamo soltanto alla lentezza dell'amministrazione giudiziaria

condizioni delle carceri nel nostro Paese, condizioni che, in tante situazioni e sotto molti aspetti, assumono ancora il carattere di una violazione sistematica dei diritti umani.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, la scelta di istituire una Commissione speciale per i diritti umani è un segnale importante dell'impegno assunto dal nostro Paese su un tema tanto delicato. Spero anche che tale scelta sia propedeutica a rendere questo tipo di Commissione una Commissione permanente nella vita del Senato. Ancora oggi, troppo spesso, la distanza tra le alte parole contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la realtà di troppe parti del mondo è drammatica e abissale. «Ogni individuo ha diritto alla vita e alla sicurezza», recita il testo della Dichiarazione. Come suonano lontane e flebili tali parole se pensiamo alle condizioni di vita in Darfur o nel Corno d'Africa, realtà dominate dai signori della guerra. la scelta di varare la Commissione speciale deve essere compiuta da quest'Aula nella consapevolezza del grande impegno che ci aspetta. Oggi parlare di diritti umani, nonostante alcuni passi avanti compiuti nel corso degli anni '90, è forse più difficile di ieri. ieri. Non possiamo non riconoscere come l'istituzione del Tribunale penale internazionale e del Consiglio per i diritti umani dell'ONU siano stati passaggi importanti, strumenti che devono far guardare con ottimismo al futuro di un mondo più equo e giusto. Ma accanto a questi passaggi positivi non possiamo non avere la consapevolezza della drammaticità della situazione che abbiamo intorno. Il ritorno in campo della guerra, dopo cinquant'anni di pace, di guerra «calda», fatta di corpi dilaniati e di bombe, è un dato che non possiamo non porre alla nostra attenzione. Una guerra spesso definita preventiva e permanente, dove i dritti concreti e materiali delle donne e degli uomini sono la prima vittima in qualunque realtà. Non possiamo non notare come tanti, tantissimi richiami che una associazione come Amnesty International ricorda alle nostre coscienze con il suo rapporto sui diritti umani, sono legati alla situazione di conflitto che viviamo anche qui, nel nostro Paese. Sarebbe banale ricordare Guantanamo ed elencare a quanti articoli della Dichiarazione universale quella struttura contravviene. Il punto, deve essere chiaro, non è un presunto anti-americanismo. E' invece la convinzione che è proprio nei momenti di difficoltà che la democrazia deve dimostrare la propria forza, garantendo il rispetto granitico dei propri princìpi. E questo non è avvenuto. Ecco, questo è un passaggio determinante della nostra riflessione: la guerra non è una soluzione, ma è una parte del problema. Vediamo quotidianamente come di fronte alla negazione dei diritti umani la guerra non sia una risposta, come l'opzione militare di «esportare la democrazia» sia non solo una ipotesi estremamente arrogante, ma sia una ipotesi dalle conseguenze drammatiche sul corpo vivo della società. In maniera davvero laica e opposta a qualunque pregiudizio dovremmo interrogarci degli effetti profondi della guerra in Iraq e di quel drammatico bollettino da guerra civile, che quotidianamente appare sui giornali sempre più distratti. Noi non possiamo accettare una Commissione che sia un lavacro delle coscienze: serve indagare perché in troppi Paesi del mondo la pacifica convivenza delle persone è messa continuamente e drammaticamente a repentaglio. Serve indagare, cercare di capire, approfondire, ma poi serve anche agire, con uno scatto di volontà. «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura»: questo dice l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. E allora noi senatori abbiamo un modo chiaro di dimostrare come quello di oggi non sia un dibattito di anime belle, un voto per poi dimenticare e passare ad altro. La rapida approvazione, anche in questo ramo del Parlamento della legge che introduce il reato di tortura nel nostro ordinamento, a 59 anni dall'approvazione della Dichiarazione universale, sarebbe un gesto, seppur tardivo, molto, molto importante. Così come sarebbe finalmente importante non far dipendere il tema dei diritti umani dalle convenienze economiche o geostrategiche. Troppi nostri prioritari *partner* commerciali sono Paesi, nella valutazione di tutti gli organi indipendenti internazionali, in fondo alle classifiche in materia di rispetto dei diritti dei loro dei loro cittadini. E allora io spero che nel nostro Paese e in tutte le istituzioni cresca la consapevolezza che, accanto alla bilancia commerciale tra i Paesi, ci sono altri parametri altrettanto se non più importanti del denaro e del profitto. cinquanta anni non siamo riusciti a rendere queste norme basilari, questi diritti inalienabili, un patrimonio dell'umanità. E già crescono intorno a noi nuove domande, nuovi bisogni, nuovi diritti che chiedono di essere accolti. Basti pensare alle evoluzioni della comunicazione e dell'informazione: con drammatica frequenza, in parti diverse del mondo, vengono imprigionati non solo giornalisti, ma anche semplici cittadini che hanno deciso di raccontare, attraverso le nuove tecnologie, la repressione e le umiliazioni di tante dittature. Le opportunità moderne della comunicazione incattiviscono il potere e noi dobbiamo essere vigili, senza pensare che questi nuovi conflitti tra potere e libertà siano conflitti di serie B. Oppure penso al diritto ad un ambiente sano, non asservito a logiche di profitto, non massacrato e cementificato. Forse questo è un diritto non solo nostro, ma anche delle generazioni future. Serve insomma un lavoro umile e di lunga lena, che rifugga dall'arroganza dei primi della classe, anche perché dobbiamo avere la consapevolezza che primi della classe, purtroppo non siamo. Cito alcuni elementi che dovranno essere al centro della nostra iniziativa: penso alla necessità di un centro indipendente. Il 28 ottobre 2005 il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, in risposta al rapporto presentato dall'Italia sull'applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha raccomandato la creazione di un organismo nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani. Su questo non possiamo che registrare un ritardo, visto che in questa fase siamo ancora al dibattito in Commissione alla Camera. E poi, ancora, le note vicende delle operazioni segrete con cui persone sospettate di terrorismo sono state trasferite dal nostro verso altri Paesi, al di fuori di qualsiasi procedura o supervisione giudiziaria, segnano anche qui, in Italia gli effetti devastanti del clima di guerra a cui facevo prima riferimento. Infine, credo che ci sia un elemento che non possiamo sottacere se ci interroghiamo della qualità del rispetto dei diritti umani basilari nel nostro Paese: mi riferisco alla condizione di vita dei migranti, di quegli uomini che spesso scappano dalla povertà, dalla fame, dalla guerra e tra questi, soprattutto i minori, i ragazzi. Ogni anno centinaia di minori arrivano in Italia attraversando il Mediterraneo su piccole barche insicure, insieme a più ampi gruppi di adulti, in fuga dalla violenza e dalla povertà. Dopo l'arrivo, il nostro Paese li tiene molti giorni nei CPT, in spregio alle norme internazionali, per le quali la detenzione dei minori è una misura eccezionale da applicare solo in casi estremi. Un ulteriore rischio colpisce i ragazzi soli dall'età incerta: quello di essere trattati come adulti e di essere detenuti ed espulsi illegalmente, in spregio degli *standard* internazionali, i quali richiedono che, nel dubbio, essi vengano trattati come minori. I CPT sono un buco nero della democrazia, dove persone che non si sono macchiate di alcun reato vengono private della libertà personale, ma, quando si tratta di bambini e minori, i CPT sono soprattutto un'infamia inaccettabile. Un'infamia inaccettabile, perché, se davvero vogliamo costruire un mondo più equo è proprio da loro, dai bambini, dalle loro speranze e dai loro sogni che dobbiamo partire. Penso, anche in questo caso, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e a quello che ne è l'articolo più disatteso, quello che dovrebbe assicurare il diritto all'istruzione a tutte e a tutti. C'è in questa affermazione, nell'idea di gratuità della scuola richiamata in quell'articolo, quella idea grande che il sapere, la conoscenza sono sinonimo di libertà; «La scuola deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace» queste sono le parole della Dichiarazione: un impegno grande, enorme. Penso allora alla nostra scuola, non alle scuole polverose di alcuni Paesi africani, ma al nostro impegno affinché anche le nostre siano scuole di pace. Tutto questo ci racconta come sia necessaria la Commissione che spero approveremo, ma come ci serva un lavoro profondo e intelligente. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, grazie, senatore Andreotti, per la sua proposta, che anch'io sottoscrivo. I diritti umani universali, i diritti inviolabili della persona, di ogni persona, sono il tesoro più grande dell'intero cammino dell'umanità, ciò che resta dopo secoli e secoli di storia. Sono la misura del presente dell'umanità, sono la fonte del suo futuro, non ve ne è altra. Un tesoro costato prezzi altissimi. La storia è il racconto dell'orrore di ciò che siamo stati, dei diritti della persona che abbiamo violato. Violenze, guerre, razzismo, colonialismo, totalitarismi, la *Shoah*, discriminazioni culturali, etniche, sociali, sessuali, la schiavitù, la tortura, la tratta degli esseri umani e degli organi, le pulizie etniche, gli stupri, la criminalità organizzata sono l'altra faccia. Ma la storia è anche la narrazione di ciò di fronte a cui abbiamo resistito, le lotte di liberazione che ci hanno rigenerato in nome dei diritti umani e le tante azioni di umanità, di sostegno dei diritti umani nel mondo. Quei diritti Quei diritti sono oggi scritti nella Carta costituzionale, sono nelle Carte dell'ONU, sono nei Trattati dell'Unione Europea, speriamo presto nella Costituzione europea. Ma noi possiamo aspirare ad una legge fondamentale e globale, la carta della politica che noi vogliamo costruire. È ben giusto che l'Italia, la Repubblica, le sue istituzioni se ne facciano carico con la costituzione della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani, che prepari la Commissione permanente indipendente dei diritti umani, come raccomandato dall'Assemblea generale dell'ONU, con compiti di tutela e di promozione. Penso alla promozione anche sul piano culturale del Paese. L'Italia, è stato detto, è la culla del diritto, ma la nostra coscienza collettiva deve crescere molto su questo versante. E poi la Commissione deve guardare alla scuola, perché lì si costruiscono i cittadini di domani e i diritti dell'uomo sono il fondamento della cittadinanza. I ragazzi devono essere chiamati ad interrogarsi su chi è la persona, chi è l'altro, quale rispetto si deve all'altro e come deve essere la convivenza fondata sui diritti umani universali. Vi è in questo un'emergenza educativa. Posso dire che lo statuto culturale e civile della scuola è su questo tema. La Commissione dovrà ben declinare i diritti umani, i diritti delle persone, perché entrino nella cultura politica diffusa, anche del Parlamento e del Governo,

il diritto alla vita, con la doverosa presa di posizione straordinaria dell'Italia nel mondo, affinché venga cancellata la pena di morte. Ma ricordo anche il diritto all'ambiente, il rispetto dell'identità, il diritto all'espressione della libertà, compresa la libertà religiosa. Bisogna inoltre cominciare a considerare le persone da quando nascono a quando crescono. il grande tema dei diritti dell'infanzia abbandonata, violata, sfruttata e mandata a fare la guerra, dell'infanzia negata nei suoi sogni e nelle sue possibilità.

delle donne di ogni condizione, delle casalinghe e delle *first lady*, delle badanti e delle donne che ovunque sono impegnate nella costruzione sociale delle nostre società. Il diritto delle donne vuol dire «no» alle discriminazioni, vuol dire coniugare le identità culturali, etniche e religiose differenti con i diritti. Abbiamo cominciato ad affrontare questo grande tema, per nulla risolto

e la costruzione delle nostre società passa anche attraverso la costruzione di diritti condivisi sulla dignità delle donne e sull'espressione del loro valore. Abbiamo bisogno di sapere che ormai i diritti sono globali, la rete è mondiale e per noi sono indivisibili, qui come in altri Paesi, in Italia come in Cina.

che è premio Nobel per la pace ed è agli arresti domiciliari da molti anni. Come può accadere questo, cioè che tutto sia subordinato agli interessi, comprensibili ma non sufficienti per giustificare l'assenza di questi diritti? Il mondo è qui da noi e noi siamo là, tutto ci riguarda: il mondo dei grandi sconvolgimenti determinati dalle migrazioni e il mondo di chi chiede asilo in nome dei diritti umani. molto importante, nella mozione che è stata presentata, l'apertura alla società civile, alle organizzazioni non governative, alle associazioni, agli enti locali e agli stessi rapporti con università e ricerca, perché ci dice che tutti siamo coinvolti in questo Ecco, signor Presidente, il segno della civiltà che vogliamo e per la quale ci impegniamo: la civiltà delle persone, del diritto che tutela i diritti, la civiltà in fondo della pace, del bene comune e della giustizia. Allora, penso anch'io che l'azione della Commissione debba essere volta molto a influire sul piano internazionale e sul piano interno con una sorta di saldatura fortissima tra politica estera e politica interna, ma anche ad essere punto di riferimento di una nuova forte crescita culturale e democratica dell'Italia, che fortemente, anche con questo impegno, oggi ed in questa sede

Presidente, college e colleghi, il senatore Martone ha firmato fin dall'inizio la mozione presentata dal senatore Andreotti, che perciò integralmente approviamo e appoggiamo. Mi limiterò pertanto ad illustrare due o tre argomenti sui quali ci piacerebbe che la Commissione iniziasse e stabilisse i suoi lavori, non senza però aver detto che l'unanime e appassionata adesione di tutto il Senato alla mozione del senatore Andreotti dimostra *ad abundantiam* l'utilità dei senatori a vita

e luxemburghiana. Voglio vedere chi sostiene che non ho il diritto di esserlo e che magari me ne dovrei anche vergognare; me ne glorio, invece, alla faccia di tutti. Intendo

dieci anni dopo che a Nairobi non si era riusciti ad arrivare ad una conclusione, siamo riuscite - c'era anch'io perciò posso dire «siamo» - a stabilire unanimemente il principio secondo cui l'integrità fisica è bene non disponibile. Questo Questo elemento, ripreso nel nostro ordinamento, ci consentirebbe di dare una tutela alle donne islamiche che eventualmente volessero nel nostro Paese essere garantite nella loro integrità fisica rispetto a quella pratica che non ha niente a che fare con il corano, com'è come è stato stabilito in dieci anni di ricerca.

citiamo il popolo dei curdi a titolo simbolico per ricomprendere qualsiasi altra identità culturale, nazionale oppressa o negata. C'è un altro punto sul quale ci piacerebbe attirare l'attenzione: una convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone portatrici di *handicap*. Questo è un elemento che a noi sembra di dover particolarmente sottolineare perché addirittura - e in proposito la Commissione avrebbe una funzione politica politica di tipo quasi costituzionale - ci sembrerebbe quasi che da questa definizione sarebbe possibile ricostituire uno Stato sociale - una delle glorie dell'Europa, ma ormai cancellata - a fondamento non lavorista, ma umano, comprensivo

Da quello che loro mi dicono, la possibilità di avere canali formativi, la possibilità di sviluppare ricerca scientifica, di sviluppare addirittura delle nuove professionalità, aprirebbe dei grandi orizzonti. Non dobbiamo pensare ai portatori di *handicap* soltanto come a persone menomate: spesso sono persone che, semplicemente, noi non mettiamo in condizione di incontrare i codici conoscitivi che servirebbero loro. Il caso dei dislessici, da questo punto di vista, è eloquentissimo. Mi scrive una logopedista, madre di un dislessico, che è diventata un'eccellente logopedista proprio per curare suo figlio. È del tutto fuori dai canali dei normali istituti del lavoro e, tuttavia, lei ha una grande professionalità che esercita nei confronti di suo figlio e per l'associazione. Ma quante associazioni possono fruire di ricchezze di questo genere? C'è una disparità anche nella società civile. Se noi potessimo mettere nel diritto e nei diritti esigibili la possibilità di avere accesso agli strumenti conoscitivi, credo ne avremmo un vantaggio generale. A me, che sono molto anziana, interesserebbe sapere se qualcuno ha studiato per i giovani che ci possono essere delle interruzioni tra il pensare, il parlare e lo scrivere, me ne servirei anch'io all'occorrenza.

Il lavoro di questa Commissione si presenta come un lavoro di continuità rispetto a quanto già svolto nella passata legislatura e in quella precedente, anche come un lavoro che si coniuga con tutto quello che il Ministero degli esteri ha svolto nel recente passato, che è sempre stato improntato ad una difesa forte, chiara ed inequivocabile dei diritti umani. Potremmo definire i diritti umani come dei passi nel deserto, dei passi leggeri, impalpabili, che attendono la collaborazione degli uomini per fare dell'oasi la normalità; un deserto che è fatto di dune, delle dune a volte insormontabili che hanno visto tante persone, intere popolazioni private della vita, del cibo, dell'acqua, ma anche dell'istruzione e, purtroppo, dei diritti politici e civili. Tutti questi diritti sono stati negati, alcune volte insieme, altre volte come diritto particolare, individuale.

affinché questi diritti venissero scritti, riconosciuti e resi riconoscibili dentro la storia dell'umanità, ci sono voluti due conflitti mondiali. Potremmo dire che la storia dei diritti umani è ancora in corso; io la definirei la vera grande sfida del terzo millennio e anche l'utopia della speranza. Per scrivere nella storia politica di oggi una pagina di speranza dobbiamo lavorare e pensare scelte politiche che concretizzino due termini - è un po' questo il mandato che mi permetto di suggerire alla Commissione speciale sui diritti umani -: dignità e tolleranza.

per alcuni aspetti, antesignana di un lavoro che oggi il Governo, così come ha fatto anche in passato, sta portando avanti.

qui, oggi, anche l'Assemblea del Senato debba ribadire un impegno in questo senso, proprio come un mandato specifico da dare alla nostra Commissione.

necessario riconoscere che non ci sono solo i diritti umani negati; ci sono anche quelli non conosciuti. Ci sono quelli conosciuti, a noi noti, ma ci sono purtroppo anche quelli non conosciuti. Voglio portare un esempio per far capire a cosa mi riferisco. Sono stata al confine tra Haiti e la Repubblica Dominicana ed ho visto, con i miei occhi, dei bambini in carne ed ossa,

nella storia dell'umanità, perché non sono stati registrati all'anagrafe alla loro nascita. Quello è un diritto umano negato, anche un diritto umano non conosciuto o troppo poco conosciuto. Il nostro compito, il nostro mandato come Commissione, è allora quello di far emergere soprattutto quei diritti negati e non conosciuti, perché non è possibile fare una graduatoria di priorità all'interno dei diritti umani. Sono tutti diritti esigibili, diritti riconoscibili, diritti che vanno difesi, sui quali ci si deve battere e ci si deve impegnare. Credo allora che proprio in questa nostra storia italiana, ma anche europea fortunatamente (non siamo soli in questo cammino di speranza), noi vogliamo ribadire il nostro impegno forte ed inequivocabile affinché le tante verità nascoste non vengano più nascoste, ma emergano, e si impegnino non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma tanti paesi insieme, affinché quelle persone che oggi pensano di non avere voce e di non avere diritti possano scoprire che almeno alcuni di questi diritti vengono loro riconosciuti. Un attenzione particolare - la ricordavano anche alcune colleghe - credo che debba essere riservata ai diritti dei bambini e ai diritti delle donne, non come due categorie, ma come due realtà espressive della persona umana, sulle quali vengono esercitate le maggiori violenze, le maggiori negazioni. Credo che proprio a loro dobbiamo rivolgere la nostra attenzione (l'abbiamo fatto con con alcune leggi che valgono nel nostro Paese). Dobbiamo cercare di portare questo afflato di libertà, di democrazia, ma anche di fraternità all'interno della politica del mondo. Voglio concludere dicendo che il tema dei diritti umani fa emergere un linguaggio ricco di significati, importanti soprattutto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista etico; un linguaggio impegnativo (lo testimonia l'importanza che sta assumendo, all'interno dell'Unione Europea e all'interno della nostra politica nazionale). C'è quindi ancora bisogno - con la scelta di oggi lo stiamo dicendo tutti ed è significativo e positivo che ci sia una unanimità di consensi - che la Commissione diritti umani continui il percorso intrapreso e sia capace di far crescere un robusto sapere dei diritti, che veda i vari ambiti conoscitivi connessi in un processo di concentrazione sulla dignità della persona: i saperi della filosofia, del diritto, della sociologia e dell'economia (che tante volte nega i diritti), ma anche i saperi della teologia sono chiamati ad interagire efficacemente con la politica, lasciandosi coinvolgere in una sfida oggi sempre più impellente. Attraverso il lavoro paziente ma autorevole della Commissione del Senato, possiamo davvero dare un senso di speranza a chi pensa di essere dimenticato dall'umanità, ma anche a noi stessi, come afflato verso l'umanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, si è avviato, all'indomani delle tragedie della Seconda guerra mondiale, un percorso volto ad individuare una piattaforma incomprimibile di diritti fondamentali della persona. Credo sia opportuno rammentare questi diritti diritti all'Assemblea perché in qualche modo ciò che stiamo dicendo e che è finalizzato sicuramente ad un nobile scopo, quello di dare un senso alle preoccupazioni che ciascuno di noi ha per la difesa di questi inalienabili diritti, possa essere ancor più mirato negli obiettivi che persegue. Il nocciolo duro dei cosiddetti diritti umani è costituito dal diritto alla vita, dal divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani, della schiavitù e dell'assoggettamento in servitù, oltre che dal principio di legalità e non retroattività della legge. Questo è - ripeto - il nocciolo duro della piattaforma che dobbiamo ritenere incomprimibile e al tempo stesso irrinunziabile. Si tratta di un percorso che nel corso degli anni ha visto una sempre maggiore convergenza a livello internazionale. A quella Dichiarazione, infatti, hanno poi fatto seguito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1960, la Convenzione americana relativa ai diritti umani del 1969, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, i Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo del 1985, per concludere con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo del 1989. È un percorso che la Commissione che ci accingiamo ad istituire può contribuire a rendere ancora più significativo, purché questo cammino sia compiuto con assoluta onestà intellettuale e di approccio, senza strabismi né dialettici, né politici, né tanto meno di parte. In tutti gli interventi che ho ascoltato, alcuni anche calati nel contesto di specifiche situazioni, non ho sentito - e mi rivolgo in questo caso in particolare ai colleghi dell'attuale maggioranza e soprattutto a coloro che militano a sinistra di quella maggioranza - alcun riferimento a Paesi in cui palesemente anche questo nocciolo duro, quello incomprimibile, quello che non può essere oggetto di sospensione neppure in virtù di situazioni particolari, proprio per quanto a livello internazionale si è ritenuto essere comunque necessariamente tutelabile, è quotidianamente e sistematicamente violato: la Cina, la Corea del Nord, Cuba. Forse sarebbe bene ricordare anche queste realtà, cui quotidianamente assistiamo ad una sistematica violazione e frantumazione di questo nocciolo duro. Onorevoli colleghi, credetemi, chi vi parla non vuol fare sconti a nessuno. che questo percorso ha già, in questo ramo del Parlamento, una traccia preziosa, quella del lavoro della Commissione per la tutela dei diritti umani, che, sotto la guida equilibrata e sapiente del collega Pianetta (al quale credo debba essere, da questo punto di vista, tributato un riconoscimento per come ha condotto nei cinque anni precedenti i lavori della Commissione che presiede), senza misconoscere alcuna realtà, guardando anche a sistemi giudiziari di Paesi che appartengono, per quello che noi siamo abituati a sostenere, al novero dei Paesi civili, ma che pure, all'interno dei loro sistemi giudiziari o delle loro strutture sociali, annidano sacche che in qualche modo incidono su ciò che attiene all'inalienabile diritto, che ciascun uomo ha, a vedere rispettata questa incomprimibile piattaforma, a partire dal sistema giudiziario e penitenziario degli stessi Stati Uniti d'America. Dico che si tratta di una traccia preziosa perché,

che portò la Commissione ad un interessante e proficuo ciclo di audizioni e ad una serie di missioni mirate, volte a verificare cosa accadesse in Paesi ad alto rischio. Si fece soprattutto riferimento a una delle più vergognose pratiche che tuttora purtroppo caratterizza il consorzio umano, cioè la tratta, a vari livelli, degli esseri umani e, al tempo stesso, alla sistematica violazione dei diritti dei minori, sia laddove non esistono scenari di guerra e, quindi, il rispetto dei diritti umani si deve comunque innestare

esistendo questi conflitti, era necessario ancor di più verificare che questa piattaforma minima fosse comunque salvaguardata.

gli organismi internazionali di tipo istituzionale sono in grado di poter verificare e vagliare le singole situazioni che caratterizzano diverse realtà e che può anche essere opportuno affiancar loro altri organismi, alcuni a base volontaristica e altri di natura istituzionale, quale quello su cui il Senato oggi si accinge a votare.

bisogna neanche dimenticare mai che non è una partita a scadere, quindi dobbiamo avere la consapevolezza che non può essere considerata un fatto circostanziale. Pertanto, se vogliamo che questo organismo possa realmente produrre effetti nel tempo

al di là di qualunque visione di parte - ripeto che essa non può essere viziata da alcuno strabismo. Allora forse - e nel dire questo desidero riprendere e fare mie le parole del collega Strano

che il 10 febbraio a Basovizza il Senato fosse presente a ricordare un momento che ha visto quello zoccolo duro, quella piattaforma incomprimibile dei diritti umani barbaramente calpestata, non perché si tratta di nostri connazionali,

Signor Presidente, il tema dei diritti umani è centrale in una società globalizzata, perché prescinde dalla fede politica e religiosa di ciascuno per richiamarsi a principi etici universali. Il tema dei diritti umani tocca tutti gli aspetti irrinunciabili della vita dell'uomo e della sua dignità, tant'è che qualcuno li ha definiti, in maniera molto efficace e condivisibile, i dividendi della globalizzazione. Questa Commissione, signor Presidente, vuol dare un contributo alla soluzione dei grandi problemi collegati alla violazione dei diritti umani, ponendosi nel solco di una tradizione cara al Senato, che già nella passata legislatura, ma ancor prima nella XIII, avevo avuto un ruolo fondamentale sia per il collegamento sistematico con tutte le organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti umani, sia per l'essenziale funzione di stimolo per l'abolizione della pena di morte. Sempre di più ormai si sta affermando una sorta di sistema di tutela internazionale dei diritti, che si impone come comune denominatore all'attenzione anche di quei Paesi che non sono in grado di sostenerli. Penso però che ci siano ancora esempi di palesi violazioni della dignità della donna, di gravi limitazioni della libertà personale, specie nei Paesi i cui ordinamenti statuali sono ispirati al fondamentalismo islamico. Ma penso anche al fenomeno aberrante della riduzione in schiavitù delle donne, che è un fenomeno che si configura anche nell'ambito di società occidentali, considerato dalle convenzioni internazionali la prima emergenza di carattere sociale; si tratta quindi di un grido di allarme per l'umanità. Mi riferisco anche alla situazione di Cuba, dove ci sono esecuzioni capitali senza processi, dove è impedita perfino la libertà di pensiero. Ricordiamo tutti la carcerazione del nostro giornalista del «Corriere della Sera» Battistini. Penso alla pena di morte anche per reati minori in Cina; penso al fenomeno dell'infanzia abbandonata e spesso soppressa nell'America Latina; penso a sistemi carcerari degradati in più Paesi, a volte anche in Paesi democratici; penso allo sfruttamento nel mondo del lavoro, anche minorile. Signor Presidente, non possiamo restare a guardare, ma non possiamo neppure fare distinzioni nella difesa dei diritti umani, nella difesa della libertà e nella difesa della democrazia. Non ci possono essere Stati più degni di altri di tutela; la politica non c'entra con la dignità delle persone. Non si può dire mai che i diritti umani, la libertà e la democrazia vadano tutelati e siano difesi in Afghanistan e non in Iraq, perché i diritti umani non si distinguono con gradazioni, ma si difendono sempre e comunque, senza «se» e senza «ma». Non possiamo, quindi, essere testimoni passivi delle deviazioni che colpiscono l'umanità e che penalizzano soprattutto le categorie più deboli. Le nostre coscienze, signor Presidente, si ribellano. Noi vogliamo essere protagonisti della nostra storia ed è per questo che vogliamo sottolineare, anche attraverso un'investitura istituzionale e attraverso la costituzione di una Commissione *ad hoc*, l'importanza della salvaguardia dei diritti umani. Ciò conferirà al nostro Paese - ne sono certa - un ruolo ancora più incisivo nei rapporti tra gli Stati e tra i popoli, e quindi un ruolo più importante nelle relazioni internazionali, in vista dell'affermazione di imprescindibili istanze democratiche sulle quali solo si può costituire e costruire una società libera.

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti»; «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona»; «nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù»; «nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti»; «nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato»; «ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica»; «ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti»; «ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione»; «ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago (...)»; «ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute (...)»; «ogni individuo ha diritto all'istruzione Sono solo alcuni dei diritti contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: il prossimo anno ricorreranno

ancora gran parte di tali diritti siano violati in molte parti del mondo, non siano riconosciuti. Ieri è stata celebrata la Giornata mondiale di lotta contro le mutilazioni genitali femminili: 3 milioni di donne e bambine sono vittime di mutilazioni genitali. L'UNICEF stima che siano state circa 140 milioni le ragazze e le donne nel mondo sottoposte a questa usanza.

affinché quei diritti, riconosciuti all'indomani della Seconda guerra mondiale e degli orrori che ha comportato, divengano realtà praticata per l'intera umanità. Da allora si sono moltiplicate le Convenzioni e i Trattati, gli strumenti concreti di cui la comunità internazionale e i singoli Paesi si sono dotati: penso alla Convenzione sulla tortura, a quella che ha istituito il Tribunale penale internazionale

parole: «Lungi dall'essere una tragica reliquia delle sporche guerre del passato, questa pratica vergognosa persiste in ogni Continente. Il nuovo Trattato colma un vuoto nei diritti umani internazionali, proibendo esplicitamente le sparizioni forzate».

deputati ed è ora all'esame del Senato. Siamo in ritardo - unico Paese europeo - con una legge organica sul diritto d'asilo, che pure era presente

Siamo stati altresì il Paese che ha dato il via al Tribunale penale internazionale, che ha lavorato perché esso divenisse una realtà. Alla Camera è in corso, proprio in queste ore, l'esame di un disegno di legge per l'istituzione di un organismo autonomo per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, colmando anche sotto ritardo che il nostro Paese aveva cumulato. È quindi evidente che che ci troviamo di fronte alla necessità di fare quanto è possibile, in Parlamento e nel Paese, perché si proceda speditamente nella tutela, nella promozione e nella salvaguardia dei diritti umani. Da questo punto di vista, il Senato è stato il ramo del Parlamento che per primo, e con maggiore lungimiranza, ha lavorato in questa direzione. Lo ha fatto nel corso della XIII legislatura, attraverso l'istituzione di un Comitato contro la pena di morte, presieduto dalla vice presidente Ersilia Salvato, che ha svolto un'attività molto importante. proseguito, andando oltre, mantenendo il nucleo essenziale del lavoro per l'abolizione della pena di morte che ha portato, ad oggi, a un rinnovato impegno del nostro Governo e del nostro Paese per la richiesta di una moratoria universale delle esecuzioni capitali

in Italia e all'estero, affrontando i temi che stanno a cuore a tante realtà associative, a tante esperienze impegnate nella tutela dei diritti umani. Procedendo in che il Senato della Repubblica e, attraverso di esso, tutto il Paese, sia nuovamente, e con ancora maggior forza, impegnato nella tutela e nella promozione dei diritti umani in Italia e nel mondo.

estremamente ricco di contributi, di riflessioni, di idee molto concrete che saranno, e sono, il migliore auspicio che questo Parlamento può offrire all'avvio di una Commissione speciale,

legislatura, abbia creato, con il Comitato contro la pena di morte, un primo momento di presenza forte e importante su un tema fondamentale di tutela dei diritti

un mondo sempre più globale e interdipendente, Paesi democratici ed evoluti accettano limitazioni della propria sovranità, accettano cioè che autorità superiori indipendenti

dei diritti umani a casa nostra. Ciò comporta non soltanto un'azione internazionale di tutela dei diritti umani, ma anche un'azione forte, intelligente, concreta di tutela dei diritti umani sul nostro territorio. Presso la Farnesina è istituito il Comitato interministeriale sui diritti umani, che ha esattamente il compito di vigilare sul rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani sul nostro territorio.

una continuità nell'azione della politica estera nei Governi succedutisi in questi anni. Oggi, noi siamo fortemente impegnati nelle Nazioni Unite, nel foro opportuno dell'Assemblea generale, per riaprire la discussione e giungere ad una risoluzione universale sulla pena di morte che porti progressivamente alla sua abolizione. Stiamo svolgendo un lavoro molto attento, che connota le nostre relazioni bilaterali nel corso di questi mesi, nell'ambito di un'intensa campagna per tentare di raggiungere

dovere, anche etico, di combattere forme di relativismo culturale. Vi sono alcuni diritti inalienabili che per noi non sono prerogativa dell'Occidente, valori che ci appartengono in modo esclusivo, ma valori universali. È stato richiamato il il tema delle nuove forme di schiavitù, dei diritti brutalmente negati della donna in molti Paesi islamici, dell'abuso della pena di morte addirittura per reati di tipo amministrativo o applicata su minori. Abbiamo il dovere anche di segnalare e di denunciare casi-Paese. È stato ricordato recentemente il caso della Birmania: purtroppo, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione da noi sottoscritta non è passata per una veto posto da alcuni Paesi.

Noi ereditiamo un'esperienza non positiva della Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite. Oggi è stata sostituita da un Consiglio per i diritti umani - peraltro l'Italia è candidata a farne parte nel prossimo biennio prossimo biennio - che ancora sconta la passata inefficacia e ancora può essere sicuramente migliorato, ma certo una Commissione come questa può fornire anche al Governo l'indirizzo utile per rendere ancora più efficace ed efficiente l'azione del nostro Governo nel Consiglio per i diritti umani.

Signor Presidente, darò anch'io il mio contributo ai tempi del nostro dibattito. Intervengo in dichiarazione di voto per esprimere, ovviamente, il voto favorevole del Gruppo dell'UDC alla costituzione di questa importante Commissione speciale, a quest'osservatorio sui diritti umani, che caratterizza non solo la grande specificità italiana e, come ricordava il rappresentante del Governo prima, una continuità in politica estera, ma anche la vocazione della iniziativa italiana nel mondo nei fori internazionali. Nel nostro intervento precedente, noi dell'UDC della iniziativa forte di diplomazia preventiva, inaugurata dal precedente Governo con l'azzeramento e la riconversione del debito alcuni progetti nel multilaterale con le Nazioni Unite, con alcune agenzie specializzate per sostenere iniziative

un progetto che andava a rivisitare le condizioni disumane cui erano sottoposti bambini, donne e anziani in quei Paesi che amiamo definire in via di sviluppo o in quei Paesi che hanno sistemi totalitari e che magari sono accettati dai nostri mercati con prodotti alle spalle dei quali vi ovviamente un diniego dei diritti umani: lavoro nero, disumano. Questa nostra iniziativa voleva anche portare alla luce, come Governo italiano, tramite le Nazioni Unite, queste grandi specificità. Non voglio parlare ovviamente dell'Agenzia per i rifugiati, che si occupa di dare delle risposte a tutti quei problemi aperti in America Latina e in tanti altri Paesi, come la Colombia, dove esistono problemi altrettanto importanti. Credo però che il valore essenziale della Commissione speciale - e concludo, signor Presidente - sia anche quello di occuparsi delle questioni di carattere nazionale, perché credo che i diritti umani non siano solo legati alla

aspetto, voglio portare all'attenzione della Presidenza - avremo modo di parlarne nella costituenda Commissione - anche tutte le politiche sul microcredito.

e proprio in quella occasione questa strada italiana al microcredito, alla microfinanza, potrà costituire, senatore Andreotti, un'occasione per far cadere una piccola goccia in più nel mare della solidarietà,

Signor Presidente, colleghi senatori, quando si chiede a noi dell'Udeur un giudizio su atti concernenti i diritti umani, motore primo del nostro agire politico, senz'altro si sa di poter contare su un appoggio incondizionato, perché sicuramente siamo pronti a dare risposte positive a chi cerca di migliorare le condizioni della persona. L'istituzione di questa Commissione, peraltro già collaudata dalla passata legislatura, risponde ad una generale esigenza di salvaguardare e tutelare i diritti umani fondamentali, primo fra tutti tutti quello alla vita e ad un'esistenza dignitosa, condannando ogni forma di discriminazione basata su questioni di sesso, razza, religione, etnia. Infatti, grazie all'attività di raccordo con le istituzioni internazionali, si potranno creare le premesse per dare completa attuazione alla nostra Carta costituzionale, imperativa quando impone la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Questa mozione è in ottemperanza al monito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha imposto, anche all'Italia, di istituire una Commissione indipendente sui diritti umani. Perciò, votando positivamente questa mozione consolidiamo la responsabilità storica del Paese incanalata nella nostra tradizione secolare e soprattutto l'originaria ideologia dell'Udeur, da sempre fermo nel considerare i diritti umani prima ricchezza dell'umanità. *(Applausi dei

brevi, vorremmo però cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza di questa mozione. I diritti umani, di cui stasera siamo chiamati a discutere grazie alla mozione presentata dal presidente Andreotti, rappresentano un patrimonio troppo spesso calpestato, che necessita una maggiore tutela nelle istituzioni di tutti i Paesi del mondo. La prima affermazione dei diritti umani si ebbe con la redazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, siglata nel 1948, dopo le due catastrofiche guerre mondiali. Con quella Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai Paesi occidentali ma rivolti ai popoli del mondo intero e basati su un concetto di dignità umana universale. Tale Dichiarazione indicava agli Stati membri l'urgenza di promuovere un insieme di diritti umani, civili, economici e sociali, affermando che questi diritti sono parte delle fondamenta di libertà, giustizia e pace del mondo. Questa dichiarazione fu il primo sforzo legale internazionale, ma nonostante gli altri numerosi passi intrapresi, quello della tutela dei diritti umani e della persona resta un tema scottante, che necessita di misure concrete per la loro effettiva applicazione. Il Senato, già nelle precedenti legislature, ha affrontato questo delicato ed importante argomento, istituendo prima un Comitato contro la pena di morte e poi una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Pur se lodevoli, queste iniziative sono state limitate nel tempo, mentre è necessario, visti anche gli scenari di violenze, maltrattamenti e guerre, avere un'attenzione continua e costante. Pertanto, nel confermare la necessità di ricostituire una Commissione speciale, non posso che lodare l'iniziativa del presidente Andreotti, sempre molto sensibile a queste tematiche. e che anch'io ho firmato, propone di avviare l'*iter* per l'istituzione di una Commissione permanente. Questo organismo, proposto dal senatore a vita, è - a mio avviso - un valido strumento in grado di tutelare e promuovere costantemente i diritti fondamentali delle persone, sanciti anche dalla nostra Costituzione. Le esperienze svolte nelle due precedenti legislature hanno dimostrato infatti come questa tematica, e più in generale quella dei diritti fondamentali della persona, abbia una sua estrema complessità e richieda quindi un'attività coordinata ed organica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che rivolgere un plauso al senatore Andreotti per aver nuovamente richiamato l'attenzione di questa Assemblea, spesse volte avvitata in logoranti discussioni autoreferenziali, su una problematica che vede già in numerosi Paesi europei l'istituzione di organismi permanenti, che tra l'altro ci vengono anche raccomandati dalla stessa Assemblea generale delle Nazioni Unite.

il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che fu ratificato dalla comunità internazionale nel 1976. Questi due prodotti sono il frutto di una umanità che usciva dalla tragedia della Seconda guerra mondiale, dai cancelli di Auschwitz e dal crimine di Hiroshima e Nagasaki.

Non a caso, l'*incipit* del Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». In sostanza, il Preambolo ricorda

umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Ho voluto ricordare queste parole, perché in quegli anni si usciva finalmente da una visione eurocentrica, in cui tutto il patrimonio sui diritti e sulla irriducibilità individuale era essenzialmente occidentale, bianco, maschio e cristianocentrico. E questo è un po' il *deficit* culturale del nostro impianto giuridico in relazione al resto del mondo. Successivamente la giurisprudenza e la sensibilità dei diritti hanno portato anche il diritto di seconda, terza

In tutto questo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è parte della Costituzione che il nostro Paese ha già ratificato, credo sia uno degli eventi più importanti in questa direzione perché allarga il diritto anche queste e ad altre generazioni, riconoscendo il diritto all'informazione, all'ambiente, alla salute, alla pace e ad un'esistenza dignitosa ed equiparandoli al diritto dell'abitare, del mangiare, delle libertà d'opinione, religiose, di culto, eccetera. Dov'è il problema allora? Devo dire che ho sempre molta difficoltà in questo ultimo periodo a parlare di diritti. Da molti anni - anzi da sette o otto anni - assistiamo ad un uso della retorica dei diritti per azioni che contrastano con il diritto. Abbiamo assistito a guerre in nome dei diritti umani; abbiamo assistito a diritti variabili, addirittura abbiamo avuto i farisei alleati con la teocrazia la teocrazia saudita per liberare e portare i diritti e l'uguaglianza in altri Paesi. Il succo è che sui diritti e sulla retorica dei diritti si sta costruendo un'asimmetria del diritto per cui alcune questioni valgono solo per Paesi che più o meno che più o meno sono riconosciuti come tali, mentre sono variabili e opinabili per gli altri. Ricordo, ad esempio, il caso dell'Afghanistan, Paese che era primo nella lista nera e che, appena è diventato un nostro alleato, è divenuto un simbolo di democrazia; ricordo anche tutti i nostri alleati, o pseudo tali,

alla svelta. Il succo è questo ed è per questo che non è facile parlare di diritti. Certo, anche se salvassimo solo una persona dalle carceri cinesi o un dissidente russo già avremmo fatto molto, perché ogni persona comunque vale tutta l'umanità,

anche al fatto che le giurisprudenze valgono solo per alcuni soggetti. Credo che casi come quello del Tribunale penale internazionale, non ratificato da alcuni

stiano a dimostrare come sull'asimmetria dei diritti e sulla guerra, che ne fa fondamento nuovo, si sta costruendo un pianeta per cui il diritto diviene il diritto di colpire, il diritto alla guerra, il diritto di giudicare. giudicare. Dobbiamo stare molto attenti perché vi è l'irriducibilità individuale, di fronte alla quale anche i nostri dovrebbero, a questo punto, discutere e pensare molto quando, in nome della comunità, delle tradizioni, delle religioni di un popolo, vogliono imporre anche al singolo individuo stili di vita e costumi, perché - mi scusi, Sottosegretario - ma non sono d'accordo sul difendere la battaglia contro il relativismo culturale. É infatti proprio questa battaglia di integralismi religiosi e politici politici che costringe l'individuo ad assoggettarsi o alla comunità o alla maggioranza; ma vi è anche una dittatura della maggioranza, se non sei in grado di difendere gli stili di vita di tutti. Come Gruppo appoggiamo fortemente questa iniziativa. Riteniamo che anche solo aiutare la società civile in ogni posto, anche solo salvare singoli individui, anche entrare nelle contraddizioni, è fare cosa di cui saremmo molto orgogliosi, oltre a

che pretendono di dare e di partecipare allo sviluppo della democrazia quando non hanno assolutamente fatto i conti con loro stessi.

la Carta dei diritti dell'uomo, ciò che ha sancito la Carta europea sull'inintangibilità del corpo come tale e del soggetto come tale, è un dato di fronte al quale persino lo Stato deve fermarsi di fronte all'inviolabilità della persona umana e della sua esistenza fisica. Purtroppo, assistiamo - lo dico con molta amarezza - a cause giuste gestite per fini

ed io dico anche per il 1917, con l'emancipazione dei popoli, delle masse oppresse che hanno ritrovato nella storia una dignità che li voleva negati per diritti divini o per diritti di autorità. Credo che sui diritti ci sarà un grande lavoro. Sono disponibile, mi piace molto

curiosità di conoscenze diverse nell'uguaglianza e, tuttavia, anche nella differenza. Stiamo, però, molto attenti: oggi i diritti rischiano di essere l'arma più letale per legittimare guerre infami e riprodurre l'oppressione di sempre di questo mondo. Quindi, stiamo attenti.

quello della promozione dei diritti umani nel Paese e a livello internazionale. È un percorso nel quale - lo abbiamo visto nella scorsa legislatura - i Parlamenti possono svolgere un ruolo di primo piano attraverso gli strumenti della diplomazia parallela, popolare, della diplomazia dal basso, stimolando, anche criticamente, senza guardare in faccia a nessuno, come è stato detto, l'iniziativa del Governo e recependo le istanze e le proposte della società civile. Molti, però, sono ancora i nodi che dobbiamo contribuire a sciogliere. Molti sono stati già affrontati nel corso di questo importante e informatissimo dibattito, altri un po' meno. Il primo riguarda certamente la relazione tra interessi geopolitici e geoeconomici e promozione di diritti umani. Come diceva il collega Silvestri, spesso e volentieri, con il pretesto buono di promuovere i diritti umani, si rischia di giustificare una forma di interventismo umanitario che invece causa altre tragedie per i popoli supposti beneficiari. Il secondo nodo, che ho sentito poco però in quest'Aula, riguarda la relazione tra esigenza di assicurare la sicurezza dei cittadini, della collettività dei cittadini - un elemento, questo, cruciale nel contratto sociale tra Stato e cittadini - e, al contempo, esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani, diritti violati dalle *extraordinary* *rendition*, dalla tortura per procura, da Guantanamo e dalle legislazioni di emergenza. A casa nostra, penso ai diritti violati di Abu Omar, Kassim Britel, Maher Arar e altri malcapitati spediti e transitati a bordo di voli CIA e torturati in quanto presunti membri di Al Qaeda. alle decine di migranti espulsi in quanto presunti terroristi, spesso con il rischio di consegnarli alle patrie galere o al trattamento dei loro carcerieri. Non dimentichiamoci, infine, della tragedia del G8 di Genova. Il terzo nodo riguarda l'indivisibilità, l'universalità e l'intergenerazionalità dei diritti umani, di quel nesso imprescindibile tra diritti di varie generazioni, quelli civili e politici, ma anche quelli economici, culturali, sociali e ambientali, troppo spesso compressi in nome del libero mercato o dell'economia. Dal diritto al cibo, all'acqua, alla terra, alla casa, alla salute, all'accesso ai saperi, l'emergenza riguarda i cittadini di tutto il mondo, non solo quelli del cosiddetto Sud del mondo, giacché ormai questa vecchia distinzione tra due emisferi del Pianeta non ha più senso. Troppo spesso si tratta dei diritti umani come appendice di politica estera, quasi solo declamatoria, e si trascura un fattore essenziale, ovvero che non potrà esserci una vera affermazione dei diritti umani senza il superamento definitivo della politica dei doppi *standard*. È un problema anche etico, di etica della politica, per la quale chi governa oggi deve tenere in considerazione diritti che prescindono dalle frontiere geografiche o da quelle fissate da un concetto restrittivo e ipocrita di sovranità. Per fare ciò abbiamo bisogno anzitutto di cambiare la lente attraverso la quale valutiamo i fatti di casa nostra. Ad esempio - e ce lo dice l'ONU - i tagli ai fondi sociali e per la casa comportano una violazione di diritti umani, l'espulsione di rom o lo sfratto forzato vanno letti non come problemi di ordine pubblico, ma come violazione dei diritti umani. L'impossibilità dei diversamente abili di avere una vita degna sarà da considerare una violazione dei diritti umani, come anche la difficoltà di un cittadino di un altro Paese (che molti chiamano extracomunitario) di venire nel nostro Paese per costruirsi una vita degna. Anch'essa è una violazione di un diritto umano, quello alla mobilità. In questo scorcio di legislatura si sono compiuti importanti passi avanti verso l'adozione di una legge sulla tortura, si lavora per l'adozione di una legge organica sull'asilo politico e per la costituzione di una autorità nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani. L'Italia si sta adoperando in sostegno ad una moratoria sulla pena di morte. C'è però bisogno di un forte cambiamento di prospettiva culturale e politica nel nostro Paese, perché, a mio parere, è in questo cambiamento che si rinnova la democrazia e il rapporto tra cittadini e cittadine e chi Per far ciò sono necessari strumenti efficaci, accessibili, partecipati, che siano sentiti dalla collettività come propri, come patrimonio comune, e non come un ennesimo orpello burocratico o amministrativo. Come diceva Richard Falk, un importante attivista per i diritti umani: «È necessario un processo di internazionalizzazione dei diritti umani nella relazione tra stato e società. È lo spirito del controllo democratico che conta». Allora, e concludo, la ricostituzione della Commissione straordinaria sui diritti umani può svolgere un ruolo di grande importanza a tal riguardo, ad una condizione, essenziale: che oltre alla sostanza si dia centralità anche al processo e che si continui nel solco del lavoro svolto nella scorsa legislatura, seguendo un approccio partecipato che riconosca pienamente il ruolo di chi, nella società civile e non solo, nel nostro Paese e non solo, ha in questi anni lavorato duramente per questa sfida di civiltà, di chi oggi rischia anche la vita per questa sfida di civiltà (non noi che sediamo comodamente in questa Aula),

(detto così sembra quasi che fosse a favore della pena di morte, ma, insomma, ci intendiamo), che fu autorevolmente ed efficacemente presieduto dalla senatrice Salvato, quanto riguarda la XIV legislatura, alla Commissione speciale, altrettanto autorevolmente ed efficacemente presieduta dal collega Pianetta. Io ebbi l'avventura di essere componente dell'uno (il Comitato) e dell'altra (la Commissione). Per la verità, nel corso della XIII legislatura, ebbi anche la possibilità di occuparmene in maniera intensa; fu un'esperienza straordinariamente importante, per la mia formazione politica e per la mia formazione morale. Nella XIV Nella XIV legislatura così non è stato, perché il concomitante impegno alla Presidenza della Commissione giustizia mi ha di fatto impedito di partecipare

fonte di grande insegnamento. Ho tratto una conclusione da questi dieci anni di lavoro su questo tema da parte del Senato: in una condizione italiana, da tutti conosciuta internazionalmente, di grande conflittualità politica e, soprattutto, in una fase

in termini - se il lavoro parlamentare sarà svolto nella maniera rispettosa con cui l'ha condotto il senatore Pianetta - di complemento e di ausilio rispetto alle strategie e alle azioni di Governo in politica estera.

dell'Assemblea del Senato. Sono stato presentatore del documento n. 1 di modifica del Regolamento del Senato.

Con quel documento proponevo qualcosa di assolutamente identico, nell'obiettivo, a quanto ora è perseguito con la mozione proposta dal presidente Andreotti.

umani. Per la verità (ricordo questo episodio quasi come un aneddoto; del resto, il presidente Andreotti non me ne vorrà, lui di aneddoti ne ha consegnati moltissimi a questa Assemblea e ogni volta lo ringraziamo per la sapidità con cui lo fa), anche nella scorsa legislatura proposi una soluzione di questo tipo, che alla fine venne abbandonata per la resistenza dei colleghi che erano allora all'opposizione. I mesi successivi a quel momento mi videro più volte raggiunto dalla senatrice De Zulueta, la quale, avendo meglio

di una Commissione speciale, che oggi c'è e domani può non esservi. La politica del nostro Stato, gli interessi del nostro Parlamento e l'autorevolezza - che prima ho richiamato - che il nostro Parlamento può esprimere su questi temi sono

aspetto. Il nostro Paese vede aggiungersi popolazioni provenienti dai più diversi Stati e dalle più diverse Nazioni, con culture ed etnie differenti. Diverse sono le opinioni sul fenomeno - non è questa la sede per affrontarlo - ma si tratta di una realtà consumata quotidianamente. Dietro queste situazioni vi sono diritti forse a volte non compiutamente rispettati, anche nel nostro civilissimo Paese. Allora, in una Camera Alta, un organismo stabile, una Giunta che - ripeto ‑ una volta istituita tale rimane nel corso delle legislature e non deve essere di volta in volta ricostituita e che sia guardiano di qualcosa che è indisponibile, non negoziabile e non rinunciabile per ciascuno di noi, a me sembra essere la soluzione

*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la costruzione del sistema giuridico internazionale di protezione e di tutela dei diritti umani è tra le grandi conquiste che l'umanità ha saputo conseguire. Al perfezionamento del sistema di tutela dei diritti umani ed all'ampliamento della sfera dei diritti fruibili dai singoli individui e dalle comunità organizzate fa purtroppo da contraltare il moltiplicarsi degli episodi di violenza, di sopraffazione, di guerra e di miseria che, a livello mondiale, con il carico di contraddizioni che è in grado di generare, rischia di avere un effetto destabilizzante per i delicati equilibri dei rapporti internazionali e di rendere a dir poco evanescente ogni affermazione di principio inerente la tutela della libertà e della vita. vita. Infatti, negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi in modo drammatico della violazione dei diritti più elementari, con un aumento, specialmente negli anni Novanta, dei conflitti interetnici e delle guerre civili. Crimini aberranti come il genocidio e gli stupri etnici, che si ritenevano scomparsi dopo gli errori e le barbarie della Seconda guerra mondiale, nonché fattispecie penali ormai ritenute estinte come la riduzione in schiavitù, sono tornati tristemente d'attualità. Il terrorismo internazionale, anche dopo i terribili fatti dell'11 settembre 2001, con il suo legato di morte e di odio, rischia d'indebolire il sistema di protezione dei diritti umani nel suo complesso, non solo perché, seminando violenza, nega l'elementare rispetto della vita e della dignità delle vittime, ma anche perché alimenta un clima collettivo di insicurezza che, con il negare le libertà di alcuni, rischia di pregiudicare la dimensione universale degli stessi diritti La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha posto in concreto il principio della difesa della dignità degli esseri umani come obiettivo primario da conseguire nell'ambito delle relazioni internazionali ed oltre gli angusti spazi della sovranità dei singoli Stati. Da allora il sistema internazionale di protezione dei diritti umani si è sviluppato in modo incisivo, non solo nell'ambito privilegiato delle Nazioni Unite, ma anche attraverso la stesura di apposite convenzioni e trattati internazionali aventi carattere regionale e continentale, che hanno progressivamente esteso le categorie dei diritti e gli spazi di fruizione degli stessi. Un ruolo del tutto particolare e peculiare fra i documenti internazionali solennemente affermati spetta a quelli destinati alla tutela dell'infanzia. Tuttavia, la piaga del lavoro minorile, il traffico degli esseri umani, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, l'indisponibilità dei farmaci costituiscono tutti momenti di estrema fragilità per l'infanzia del pianeta. Ho voluto citare la tutela dell'infanzia, ma l'insieme delle carte, delle convenzioni, delle dichiarazioni, sia in ambito ONU che nelle varie organizzazioni regionali, coprono l'intera gamma degli argomenti attinenti i diritti umani.

Tutelare concretamente, promuovere i diritti umani è un dovere per ogni popolo, perché, come ha detto Benedetto XVI davanti al corpo diplomatico: «Vorrei ricordare quanto stabilito con grande chiarezza nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, vale a dire che i diritti fondamentali dell'uomo sono i medesimi sotto tutte le latitudini». Questo non è solo il riconoscimento dell'universalità dei diritti umani, ma soprattutto il riconoscimento che attraverso i diritti umani si esprime il valore unico e condiviso di ogni membro dell'umanità;

parlando dei diritti umani, ebbe a dire: «Il primo elemento è l'incondizionatezza con cui la dignità umana ed i diritti umani devono essere presentati come valori che precedono qualsiasi giurisdizione statale». Dunque, questo valore fondamentale dei diritti umani deve essere promosso e tutelato da tutti, istituzioni e società. I principi dei diritti umani, nella loro accezione più ampia, necessitano pertanto di una diffusione, di un'assimilazione e di un consolidamento. Il Parlamento italiano, con il sostegno di tutti i Gruppi parlamentari italiani - lo abbiamo visto qui questa sera dedica da tanto tempo grande attenzione ai diritti umani, ed è arrivato a condurre battaglie in nome del rispetto della dignità e della tutela di ogni essere umano. Nella XIII legislatura - è stato ricordato - si è istituito un Comitato per seguire i progressi compiuti a livello internazionale in merito all'abolizione della pena di morte. Nella XIV legislatura si è deciso di andare oltre, con l'istituzione di una Commissione straordinaria, con il proposito di osservare, studiare e prendere iniziative, anche creando contatti con le istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali e recandosi laddove, in Italia e all'estero, fosse necessario stabilire intese per la promozione e la difesa dei diritti umani. Vorrei qui ringraziare il presidente Andreotti e i colleghi per aver voluto apprezzare l'attività svolta dalla Commissione nella precedente legislatura e per essere, il presidente Andreotti, il promotore della nuova Commissione. Commissione precedente ha svolto una funzione di stimolo alla promozione e alla salvaguardia dei diritti umani ed all'affermazione di una cultura di difesa della dignità e della vita di ogni essere umano, ponendosi come momento di raccordo tra il mondo della società civile e quello istituzionale. A tale scopo, essa ha avviato una specifica indagine conoscitiva sui livelli e sui meccanismi di tutela dei diritti umani nel mondo. L'indagine ha preso le mosse dalla tesi che i diritti umani nella loro universalità rappresentano, o dovrebbero diventare, la bussola di ogni iniziativa in campo internazionale. Si è dunque andati oltre la pena di morte e sono stati molti i temi trattati. Porto come esempio il traffico degli esseri umani per l'implicazione internazionale e i risvolti anche nazionali. Si tratta di un fenomeno che prova che le violazioni di diritti umani trovano terreno fertile laddove c'è un ritardo nello sviluppo economico e sociale. Dove ci sono povertà e ignoranza il campo è libero per il pregiudizio e per il disprezzo della vita. Dunque, la tutela dei diritti umani è collegata ai problemi dello sviluppo, ovunque. La sede privilegiata in cui questa condivisione di fondo può realizzarsi sono le Nazioni Unite; il lavoro delle Nazioni Unite è fondamentale, ma purtroppo insufficiente. Ripensare le Nazioni Unite doveva essere l'impegno, ed è l'impegno fondamentale. Lo aveva detto Kofi Annan, «Se non si rinnova l'intero sistema di tutela dei diritti umani le Nazioni Unite non saranno in grado di riguadagnare la fiducia dell'opinione pubblica». Sin dal dicembre 2004 il rapporto dell'*High Level Panel* aveva lanciato l'allarme sulle grandi emergenze umanitarie del pianeta. Il quadro è ancora più allarmante se si aggiungono le insidie legate alla proliferazione di armi nucleari, radiologiche, chimiche e biologiche e le minacce alla stabilità mondiale causate dalle organizzazioni del crimine organizzato Sono problemi complessi che gli Stati da soli non possono affrontare e risolvere. Il ruolo delle Nazioni Unite è quindi indispensabile, così come è indispensabile ripensarne l'assetto e le funzioni. La riforma a metà cui si è giunti, pur rappresentando un importante passo avanti, non può essere considerata sufficiente. La creazione di un Consiglio per i diritti umani va valutata positivamente, ma ne restano indeterminate le funzioni e la struttura. Il rafforzamento delle Nazioni Unite nella capacità di intervenire in missioni di *peacekeeping* e di ricostruzione è un fatto positivo, ma occorrerà vedere come verrà attuato in concreto. Sarà dunque indispensabile in futuro accrescere gli sforzi perché nell'ambito delle Nazioni Unite si possa giungere a soluzioni condivise su problemi articolati e complessi. L'Italia in questo biennio come è già stato ricordato - fa parte del Consiglio di sicurezza ed è candidata per il Consiglio dei diritti umani. Abbiamo dunque l'opportunità di dare un significativo contributo su tali argomenti. Anche l'Europa dei 27 deve compiere ulteriori passi in avanti in materia di libertà, democrazia, uguaglianza e legalità, pluralismo, non discriminazione, giustizia, solidarietà, parità fra uomini e donne. Pertanto, sono molte le attese dell'Unione Europea. Non si può certo ancora parlare di fallimento della globalizzazione; piuttosto, preferisco parlare di globalizzazione incompiuta. Certamente, siamo purtroppo ben lontani dalla distribuzione dei dividendi della globalizzazione. Fu proprio Fu proprio il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, durante il rapporto annuale all'Assemblea generale di alcuni anni fa, ad osservare che: «La combinazione di sottosviluppo, globalizzazione e rapidità dei cambiamenti pone delle sfide particolari al regime internazionale dei diritti umani». Credo che in questa non facile cornice possa continuare a svilupparsi il lavoro della Commissione, che ci apprestiamo a istituire e per la quale Forza Italia esprime un voto favorevole, sui molti temi cui ho già accennato, con il metodo del confronto diretto con le realtà difficili in Europa e in ogni parte del mondo; di confronto diretto con i protagonisti dell'impegno umanitario e con l'impegno istituzionale e la consapevolezza di ciascuno sui gravi problemi che minacciano quotidianamente i diritti fondamentali della persona. Ecco dunque, a mio avviso, il profilo dell'attività della futura Commissione parlamentare che, in prospettiva, mi auguro possa diventare permanente. Il Senato potrà così continuare a dare il proprio contributo. per i diritti umani è stata all'estero, ovunque le nostre rappresentanze diplomatiche hanno ringraziato il Senato perché l'attenzione della Commissione consentiva loro di sottolineare il ruolo dell'Italia su argomenti così importanti e fondamentali. base dell'esperienza precedente, potrà affrontare temi generali e anche casi particolari. Voglio concludere - mi permetta, signor Presidente - riferendo un triste e terribile episodio di cui abbiamo parlato con il presidente Karzai. diritti umani non ha potuto fare nulla per Nadia Anjuman, la venticinquenne poetessa afgana uccisa a bastonate dal marito lo scorso mese di novembre, poco prima dell'arrivo della Commissione a Kabul. Nadia aveva scritto una raccolta di poesie dal titolo

di Nadia Anjuman, tratti dalla poesia «Il canto più triste»: «Sono ancora io che mi riempio di ricordi. Anche la notte, un po' alla volta, va per la sua strada e io divento il più triste canto d'addio». Sono versi che dicono della solitudine, dell'abbandono, della disperazione di chi non ha cittadinanza, non ha voce e non ha diritti. Per questo dobbiamo lavorare con impegno tutti insieme.

della democrazia - degli uomini e delle donne, nel rispetto delle loro differenze e della loro universalità (un aspetto essenziale che abbiamo scoperto) - e all'avanzamento dei nuovi diritti che in questi anni si sono generati. Dal 1948 quella Carta fondamentale è stata spesso stracciata in molte parti del mondo, ma dal 1948 nuovi diritti sono emersi e stanno emergendo all'interno di una nuova stagione. Giustamente nella mozione

il processo di globalizzazione in atto rende indispensabile riconoscere piena tutela ai diritti fondamentali della persona, affinché i diritti umani, intesi nella loro accezione più ampia, possano realmente affermarsi come «Legge dei Popoli»;

fare guerre che poi negano gli stessi diritti, in primo luogo il diritto alla vita, visti i morti che il mondo sta subendo a causa di queste guerre. Oggi abbiamo quindi bisogno di costruire insieme una nuova stagione che ridefinisca i diritti umani come diritti dei singoli,

tanta parte della popolazione mondiale, al diritto all'acqua, che diventa oggi uno dei diritti più importanti, e al diritto al cibo che è sempre stato, ed oggi lo è ancora di più, diritto fondamentale per poter sopravvivere,

al di là delle nostre concezioni, c'è un punto universale del nostro dibattito. Voglio concludere dicendo che in tal senso vi è un ruolo specifico

presa di coscienza di ciò che è stato per noi la guerra. In questo continente martoriato da guerre decennali e secolari, dopo la Seconda guerra mondiale siamo riusciti a costruire finalmente una coscienza che ha permesso a tutto l'Occidente di superare quella tragedia che aveva negato di fatto i diritti di tutti, di quei 100 milioni di morti della Seconda guerra mondiale

Comunità europea, ma abbiamo bisogno di costruire un articolato serio, che ci permetta di distinguere bene e di costruire un diritto per coloro che scappano dalla morte e vogliono vivere in maniera diversa in questo mondo. Sento pertanto il bisogno di dare con forza un'altra *chance* positiva a tutti noi, di dare a tutti la possibilità di

è quello che volevo dire. Mi sembra che questa nostra Commissione ci permetta di affrontarlo. Lo possiamo fare, abbiamo già fatto cose importanti nelle altre due legislature. Esistono gli strumenti e per farlo, per avere un confronto serio con tutte le società e con tutti i

Colleghi, il Presidente del Senato ha riferito alla Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, la disponibilità del Ministro degli affari esteri a rendere comunicazioni a breve in materia di politica estera, al fine di dare corso a quel dibattito che era stato richiesto da più forze politiche in seguito al voto di giovedì scorso. Poiché non si è registrata l'unanimità dei consensi circa la data del dibattito, il Presidente si è impegnato a compiere un'ulteriore verifica presso il Governo, rappresentando le posizioni dei diversi Gruppi,

della riunione di ieri, ha stabilito all'unanimità che domani mattina l'Assemblea non terrà seduta per consentire la convocazione dei Comitati della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per la revisione delle schede elettorali, nonché delle Commissioni permanenti per l'esame dei provvedimenti di loro competenza, con particolare riguardo ai decreti-legge in calendario. Resta confermato per domani pomeriggio il sindacato ispettivo. La prossima settimana, nel pomeriggio di martedì 13 febbraio, saranno esaminate le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 14 febbraio sarà esaminato, ove concluso dalla Commissione, il decreto-legge recante proroga di termini legislativi. Se possibile, sempre in quella settimana, sarà anche avviato l'esame del decreto-legge dì recepimento di direttive comunitarie approvato ieri dalla Camera dei deputati. I Capigruppo hanno inoltre convenuto di prevedere in una prossima seduta un dibattito sulle politiche ambientali.